nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

tanto che il nostro Gruppo era stato indotto a pensare di presentare una pregiudiziale di costituzionalità prima e a votare contro poi. Se l'obiettivo del decreto-legge era il raggiungimento di una percentuale di copertura vaccinale adeguata a raggiungere la cosiddetta immunità di gregge ed evitare quindi il rischio di contagio, non era con la coercizione per legge che si sarebbe raggiunto. Sarebbe invece stato necessario informare, comunicare e motivare le famiglie sulla necessità di vaccinare i figli per tutelare loro stessi e gli altri. Ciò è dimostrato dal fatto che è vero che su 28 Paesi dell'Unione europea 15 hanno intrapreso la strada dell'obbligatorietà sancita per legge, ma è altrettanto vero che negli altri 13 Paesi ciò non succede - guarda caso - sono quelli con la più alta percentuale di profilassi. Tra l'altro, l'obbligatorietà per decreto, supportata e giustificata da pareri il più delle volte provenienti da istituzioni e ambienti vicini e contigui al Governo, e dunque interessati,

come si può solo immaginare di segnalare alla procura dei minori genitori che, per motivi vari, non sono d'accordo su un provvedimento che riguarda direttamente la salute dei loro figli? Come si può solo immaginare che le istituzioni scolastiche e giudiziarie del nostro Paese possano sopportare l'urto di migliaia di segnalazioni e dei relativi ricorsi? Un altro punto che a nostro parere metteva in dubbio la costituzionalità del provvedimento erano le sanzioni, dell'ordine di migliaia di euro. Ciò avrebbe prodotto due categorie di famiglie, distinte e divise per censo, classe e disponibilità economica: chi poteva pagare la somma fino a euro 7.500 veniva esentato dall'obbligo, gli altri no. Ciò in un momento in cui l'ISTAT certifica che in Italia vi sono 1,6 milioni di famiglie, per complessivi 5 milioni di persone, che versano in una condizione di povertà assoluta, rendendo ancora più odiosa e inaccettabile una differenziazione degli obblighi e dei diritti basata sulla disponibilità economica delle famiglie. Da considerare, infine, il numero delle vaccinazioni. Sono un numero abnorme, alcune delle quali non giustificate da evidenze scientifiche ed epidemiologiche. Questi, in sintesi, sono i punti più controversi che ci avevano convinto dell'impossibilità di esprimere un voto favorevole. Per fortuna il percorso parlamentare, prima in Commissione e poi in Assemblea, ha profondamente modificato il testo, rendendolo più aderente alla nostra realtà e più utile a raggiungere gli obiettivi che si era prefisso, il primo dei quali è quello di informare le famiglie e aumentare la loro *compliance* verso la profilassi vaccinale. È stato cancellato l'obbrobrio della revoca della responsabilità genitoriale in caso di inadempienza; i genitori verranno invece convocati dalle aziende sanitarie e informati sulla necessità di aderire alla profilassi. Si spera che il Governo, prima ancora che questo avvenga, avvii per tempo una campagna d'informazione e sensibilizzazione, fatta nelle sedi opportune e da personale adeguato, cosa che fino ad ora è mancata. È stato ridotto il numero complessivo dei vaccini, alcuni dei quali resteranno obbligatori solo i prossimi tre anni fino a verifica e nuova valutazione clinica ed epidemiologica. Le sanzioni sono state drasticamente abbattute, in linea con le disponibilità economiche degli italiani: la nuova forbice da 100 a 500 euro di certo non risolve il dubbio di costituzionalità, ma almeno ne attenua l'impatto e le relative conseguenze sulle scelte che le famiglie potranno fare. La possibilità di praticare la profilassi vaccinale nelle farmacie alla presenza del medico è da sostenere per ottenere la più ampia copertura possibile. Si auspica, dunque, che il Governo tenga nella dovuta considerazione l'ordine del giorno presentato e accolto al riguardo. Infine, l'emendamento aggiuntivo della relatrice, che prende in considerazione la somministrazione e quindi la produzione di vaccini monovalenti e la richiesta di utilizzare vaccini sempre più puri, ha messo un altro mattone nella correzione di questo provvedimento. Tutti questi aggiustamenti hanno reso - a nostro parere - il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge molto più utile a raggiungere quello che poi è l'obiettivo: aumentare la copertura vaccinale nel nostro Paese e impedire il rischio epidemico. Ma molto resta da fare e noi saremo vigili sul prosieguo del provvedimento e su come verranno redatti e scritti i decreti attuativi. Alla luce di queste considerazioni, il Gruppo Federazione della libertà esprimerà un voto favorevole.

avrei voluto applaudire la signora Ministro alla fine dell'*iter* parlamentare di questo decreto-legge, ma purtroppo non mi sarà possibile, perché il problema dell'Italia è l'epidemia di morbillo e quindi era sufficiente a rendere obbligatoria questa vaccinazione. Io credo nell'utilità delle vaccinazioni, e proprio ieri mi è arrivata la richiesta di fare una donazione per la vaccinazione antipolio. La polio è presente ancora in tre Stati nel mondo: Afghanistan, Pakistan e Nigeria. Con soli 50 euro è possibile vaccinare 128 bambini. Pensate, se lo facessimo tutti, 38.400 bambini sarebbero vaccinati contro la polio. E lo sapete con quale vaccino? Con il Polioral, virus vivo attenuato per uso orale, come l'esempio che vi avevo fatto in discussione generale, io, semplice medico omeopata e senatore per caso. Sapete quale ditta lo produce? La Chiron di Siena, al costo di 39 centesimi per un ciclo completo per un bambino. Pensate quanti ne avremmo potuti vaccinare, al posto di assumere 20 persone al Ministero e di dare soldi tolti alla didattica ai dirigenti scolastici. Avremmo potuto salvare molte vite umane e forse eradicare definitivamente la polio. Nel bollettino della sempre citata Organizzazione mondiale della sanità leggiamo che la soglia necessaria per interrompere la trasmissione di una malattia infettiva dipende dal numero di riproduzioni di base, cioè il numero di casi secondari generati da un tipico soggetto infettato e infettante, quando il resto della popolazione è suscettibile. E il bollettino cita come fonte bibliografica il libro di Anderson e May, i cui valori sono stati riportati da molti auditi in Commissione e sono al 95 per cento solo per il morbillo. Se vogliamo attenerci alle evidenze scientifiche, occorre fornire le prove che la soglia del 95 per cento di copertura per ottenere l'immunità di gregge corrisponda a tutte le malattie infettive. Purtroppo penso che ai promotori del decreto-legge le cause sociali che hanno determinato l'abbassamento della copertura vaccinale non interessino e soprattutto non interessino le cose che più volte ho detto, lavorando sul campo e parlando da anni di questo problema con molti dei miei pazienti. La gran parte degli auditi ci ha ricordato che dobbiamo ascoltare attentamente le preoccupazioni dei genitori e lavorare con le comunità e gli operatori sanitari per creare consapevolezza, con il fine che ogni persona possa prendere decisioni consapevoli per sé e per i propri figli; il contrario di ogni genere di obbligatorietà. È estremamente importante dare informazioni basate su dati reali di benefici e sicurezza dei vaccini, cosa che non facciamo. La scienza negli anni ci ha insegnato a mettere sempre in discussione le nostre teorie ad ascoltare con maggiore attenzione proprio le ipotesi che più si discostano dalle nostre, perché è con la mente aperta a tutte le opinioni e l'animo umile che si ricerca la verità. Ho sentito più volte dire che bisogna restare in campo scientifico, ma l'impressione che ho avuto e che stiamo dando è che la scienza si sia messa al servizio, per giustificare interessi politici, economici e personali. Per fare questo si sono cancellati gli effetti collaterali dei vaccini, forse semplicemente per non dare adito a effetti contraddittori sulle vaccinazioni. Ma affermare questo vuol dire negare che ci sono persone che vivono sulla loro pelle il problema creato dalla vaccinazione, che è un qualcosa in più di una semplice punturina, come ho visto fare in televisione. È così che l'operato del medico, che dovrebbe basarsi sui principi di scienza e coscienza, si trasforma in obbedienza e accettazione di un dogma scientifico. Ho sempre difeso la pratica vaccinale e condivido il principio dell'offerta attiva e gratuita dei vaccini da parte dello Stato. Ma per quale principio scientifico dovrei costringere un mio paziente a vaccinare il proprio figlio, minacciandolo di non poter accedere al nido e alla materna, senza preoccuparmi di quanto questo pesi sotto l'aspetto sociale e psicologico sia sul genitore che sul bambino? Tutto questo per farmi sentire più sicuro che i miei figli o i miei nipoti siano protetti perché, oltre a vaccinarli, ho costretto anche gli altri a vaccinarsi. Tutto questo in nome della scienza. Anzi, se non lo faccio, sono tacciato come antiscientifico, Da quando sono arrivato in Senato, ho sentito come un mantra che dobbiamo mettere il paziente al centro della cura, prendersi cura di lui invece di curare solo la malattia, in una parola: la medicina centrata sulla persona. È quello che io, come molti medici che integrano le conoscenze scientifiche con le medicine non convenzionali, faccio tutti i giorni nel mio ambulatorio e - aggiungo - che amministratori aperti e illuminati hanno inserito all'interno di aziende ospedaliere. Se essere scienziati vuol dire non avere dubbi, vi dico che io non sono uno scienziato, ma vorrei che questo dibattito scientifico venisse ricondotto nelle sedi appropriate. Vorrei che il mondo accademico, invece di pronunciare dogmi indiscutibili, riconquistasse un atteggiamento...

Senza questo decreto, i genitori torneranno a fare i genitori, fidandosi dei propri medici e, forse, anche della politica e dei suoi rappresentanti, di cui in questo momento mi onoro di fare parte. Per tutti questi motivi, il voto mio e della componente dell'Italia

con questo decreto-legge che doveva porsi un obiettivo di sanità pubblica state spaccando il Paese e anche la comunità scientifica. Non è un decreto ragionevole, ma esagerato, forzato nelle misure, pasticciato, come è stato dimostrato in quest'Aula. È un decreto che non ascolta i genitori, quel popolo che non è contro i vaccini, ma è per la trasparenza, l'informazione e la libera scelta. È il popolo *free vax*, che cresce ogni giorno, che da settimane sta manifestando in molte piazze italiane, come quella di Roma negli ultimi giorni, e come quella di Pesaro, dove un'enorme onda arancione fatta di decine di migliaia di famiglie si è riunita, ma di cui nessun telegiornale ha parlato, nemmeno quelli della RAI. Vi parlo da padre di due bambine piccole, di otto e quattro anni, a cui ho fatto fare i vaccini, anche quelli raccomandati, vaccini di cui riconosco l'importanza.

Invece di recuperare la credibilità delle istituzioni, dicendo la verità, voi la verità la state calpestando. Questo decreto-legge è inaccettabile, perché lede la libertà di cura di milioni di minori, perché viola l'articolo 32 della Costituzione, che stabilisce che nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario, salvo in presenza di deroga che può esistere solo in stato di necessità, che oggi non c'è, Ministro, visto che anche il suo *premier* Gentiloni ha detto che non sussiste un'emergenza sanitaria nazionale. I dati epidemiologici non danno un quadro di un Paese colpito da epidemie con numeri vaccinali in caduta libera: le nostre coperture sono analoghe o addirittura superiori a quelle degli altri Paesi europei, in quindici dei quali - lo ricordo - l'obbligo dei vaccini non c'è. E poi le coperture, ancorché fossero basse, si recuperano con l'informazione *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Il Governo sostenuto dalla maggioranza sta invece tenendo un atteggiamento arrogante, perché si è inventato un stato di necessità anche con notizie false. Anche sulla salute siete ricorsi all'ennesima narrativa raccontando una vostra realtà di comodo; una narrativa destinata a crollare come quella dei migranti, secondo la quale tutti scappano dalle guerre.

i 200 decessi nell'anno successivo, quando invece i dati ufficiali del Governo britannico riportano un solo decesso nel 2013 e zero nel 2014. Da sciacalli è stata persino strumentalizzata la vicenda drammatica del bambino morto per morbillo al San Gerardo

le reazioni avverse, incluse le malattie gravi e persino le morti, quando lo stesso Ministero della salute e i tribunali riconoscono invece i risarcimenti.

di cui nessuno dovrebbe parlare. Questa, relatrice Manassero, è disinformazione e propaganda che minano il principio di sicurezza dei cittadini e che di certo contribuiscono ad aumentare la diffidenza verso i vaccini. Eppure, ci sono dei danneggiati, anche gravi: sono diverse

anni; come Giovanni Matteo, deceduto nel giugno 2016. Ho con me le lettere del Ministero della salute che lo certificano. Oppure come il piccolo Emiliano, deceduto a soli quindici mesi nel febbraio 2003. Quelli nominati sono solo alcuni dei morti documentati e riconosciuti con benefici e indennizzi dal Ministero della salute o dai tribunali italiani. degli effetti collaterali e dei danni irreversibili da vaccini è vietato parlare, perché deve prevalere il pensiero dominante, che è arrivato persino a imporre la radiazione dal proprio ordine dei medici critici verso i vaccini. punizione ha fatto persino esultare gli ipervaccinisti alla Burioni. Per voi non si deve parlare di quei vaccini che, attraverso il ricorso alle nanotecnologie, si scoprono inquinanti, con nanopolveri tossiche non biodegradabili, non biocompatibili; e non parlo solo degli adiuvanti. Questa, Ministro, non è antiscienza. È la vostra assenza di dubbi che preoccupa, come - ad esempio - sulle superficiali sperimentazioni dei vaccini, che dimostrano un'arroganza allarmante. Altro che spacciare l'obbligatorietà dei vaccini per il bene dei nostri figli e per la salute pubblica. La realtà è che la vicenda dei vaccini obbligatori è una scelta non fatta nell'interesse nazionale, ma parte da lontano. È stato deciso al Global Health Security Agenda, nel settembre 2014, a Washington, del Presidente dell'Aifa è stato deciso che per cinque anni l'Italia avrebbe guidato le strategie e le campagne vaccinali nel mondo (è scritto sul sito del suo Ministero), assecondando così - lo sottolineo - l'interesse di qualche multinazionale del farmaco, ma sulla pelle dei cittadini, anzi dei bambini, magari con la complicità di qualche dirigente del suo Ministero in palese conflitto d'interesse. Irresponsabile da parte del Governo avere prestato l'Italia come paese cavia. Questo è grave, tenuto conto che non esiste alcun Paese in Europa con 12 vaccini obbligatori, ora ridotti a 10, e non si capisce secondo quali evidenze scientifiche; numero che resta comunque alto, soprattutto se somministrati nei primi mesi di vita del bambino! In questo senso sono irresponsabili le dichiarazioni rese in televisione dal sottosegretario Faraone - che non vedo - che ha affermato: «Non credo che il fatto che l'Italia sperimenti l'obbligatorietà anche su quel numero di vaccini debba essere considerato un fatto negativo». Ma siamo matti? Siamo matti? La sperimentazione è una cosa seria e deve essere fatta su base volontaria, attraverso un consenso informato, che deve seguire un'informazione seria, completa, che faccia accrescere la credibilità delle istituzioni. Così voi state violando le norme convenzionali di medicina. Così voi le istituzioni le state affossando! Con la fase emendativa il provvedimento è stato migliorato, ma mantiene tutta la sua gravità: permangono le misure coercitive con l'obbligo di 10 vaccini e, dunque, un piano di profilassi massiva, e rimane - e questo è grave - l'esclusione dal nido e dalla scuola dell'infanzia dei bambini da zero a sei anni se non sono stati vaccinati. vaccinati. Per le scuole dell'obbligo, invece, cara senatrice Puglisi, elementari e medie, c'è invece un altro regime: qui basta pagare la sanzione, per chi può permetterselo ovviamente, creando una disparità di censo e di classe. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. No! Così non va bene! La vaccinazione non si deve imporre ai bambini ma proporre, rispettando la responsabilità genitoriale alla quale lo Stato non deve sostituirsi. Le direttrici di un serio per perseguire l'immunità di gregge dovevano passare - non attraverso un decreto-legge - da una campagna di informazione trasparente e completa, finalizzata al consenso informato sui benefici e sui possibili effetti collaterali, per consentire ai genitori di operare una scelta consapevole di adesione con convinzione alle campagne di vaccinazione; come sta facendo dal 2007 la Regione Veneto, con il presidente Zaia, che contro la vostra protervia ha già depositato il ricorso alla Corte costituzionale. È una Regione modello quella Veneta che, attraverso una corretta campagna di informazione, ha raggiunto quasi il 93 per cento di copertura vaccinale e, soprattutto, ha istituito da tempo l'Anagrafe regionale vaccinale. La Lega Nord - lo ripeto - non è contro i vaccini, ma voterà contro questo pessimo provvedimento, illiberale - e mi rivolgo ai senatori che siedono alla mia sinistra che ha nell'obbligatorietà - come definito dalla relatrice - il suo pilastro fondante, ma che per noi invece conferma l'esistenza di una dittatura del relativismo che vede il Partito Democratico uno dei principali protagonisti. *(Commenti del a sostenere milioni di famiglie per bene nella loro battaglia di civiltà e per il bene dei loro e dei nostri figli. n. 2856** Signor Presidente, onorevoli senatori, quello in discussione è un provvedimento che si inserisce nella categoria dei più delicati

partito ha lasciato liberi alcuni senatori di esprimere il loro dissenso rispetto alla posizione del Gruppo, proprio perché i principi di etica e scienza sono *border line*. Da un lato parliamo, infatti, della salute dei cittadini nel caso specifico dei nostri figli o nipoti - e, dall'altro, di una forma di educazione sanitaria che i bambini di oggi dovranno domani, una volta padri e nonni, a loro volta contribuire a diffondere. Si tratta, dunque, di un tema con tante sfaccettature che probabilmente, trasferito in un atto normativo, non convincerà mai nessuno in modo pieno e totale, a prescindere dalle legittime convinzioni di ciascuno. Date queste premesse, sarebbe stato forse preferibile procedere diversamente,

al consociativismo tra Governo, Partito Democratico/Zanda e Forza Italia/Paolo Romani, a mo' di «Colpo grosso», per citare quella famosa trasmissione

nell'approcciare al provvedimento. Il testo ha infatti subìto, sia in Commissione che nel corso del passaggio in Aula, svariate modifiche, molte delle quali

Aspetto rimarcato anche dal ministro Finocchiaro che grazie alla sua esperienza, alla sua razionalità, alla sua serietà ed alla sua preparazione è riuscita a risolvere una situazione una situazione di impasse che rischiava di far naufragare il decreto. Infatti, di fronte alla politica sanitaria del ministro Lorenzin c'è solo da mettersi le mani nei capelli.

vengono curate solo 60.000 persone, per la modica cifra di 79.000 euro a paziente (2,5 miliardi di euro in tre anni). Su questo punto specifico ricordo che Paesi come l'India sono molto più avanti di noi. A tal proposito, voglio dunque evidenziare che se

Lo ha dimostrato il Parlamento, che ha completamente stravolto il testo. La responsabilità genitoriale - argomento delicatissimo sul quale anche il mio Gruppo aveva presentato degli emendamenti nel senso delle modifiche poi apportate - non è tema da poco. Come fa un Governo a venire in Parlamento di fronte agli italiani a dire che toglie la la patria potestà? Ma come è possibile? Che "roba" usa? Sicuramente tagliata male! I minori stranieri, sia nel contesto dei flussi migratori che viviamo con sempre maggiore pressione, sia semplicemente considerando che appena lo scorso 29 marzo è stata approvata una legge su quelli non accompagnati, non è certo una questione irrisoria da poter sfuggire a un Ministro. Anche questo è un contributo che il Parlamento ha dato, stravolgendo il testo. Lo stesso numero delle vaccinazioni da rendere obbligatorie rappresenta un tassello fondamentale, alla stregua dei colloqui informativi

che non è un'invenzione, ma è parte della nostra struttura costituzionale. Ricordiamoci, infatti, che parliamo sempre di cittadini, per la loro genitorialità certamente sottoposti a responsabilità particolari, ma pur sempre cittadini che hanno il diritto di comprendere a fondo cosa stanno facendo ai loro figli e quali sono le conseguenze. Non sudditi che sulla pelle della propria prole devono esclusivamente esclusivamente sottostare alla volontà impositiva dello Stato. Non di poco conto è stata poi la decisione del Senato di di abbattere drasticamente l'ammontare delle sanzioni per i genitori inadempienti rispetto a quelle previste dal decreto-legge nella sua formulazione originaria. Il senatore Buemi, che si rifà a una tradizione socialista - ahimè - ha fatto la figura uguale

La modifica più importante, richiesta a gran voce anche dalle opposizioni ma apportata attraverso un emendamento del relatore (che ha quindi contribuito a smentire ulteriormente il ministro Lorenzin), riguarda poi la possibilità di somministrare vaccini monocomponente. Si tratta di una scelta sensata, logica e scientificamente coerente, che anche il mio Gruppo ha ritenuto di abbracciare con convinzione. Uno dei nodi molto discussi è stato poi quello relativo alla possibilità di somministrare i vaccini presso le farmacie. Questa eventualità - se Dio vuole - è stata respinta per una questione di copertura finanziaria, da un lato, e per le rimostranze di quanti, medici in prima linea, attraverso la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, hanno molto insistito sulla linea secondo la quale «l'unico luogo appropriato per la pratica vaccinale è rappresentato dalle strutture delle aziende sanitarie locali e dagli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, che costituiscono una rete più capillare e dotata di

ormai sull'onda del populismo che ha invaso la politica da tutte le parti siamo arrivati a risparmiare finanche sulla democrazia; per quanto riguarda invece l'aspetto sanitario, rimarcando che la mia professione è quella del medico, ricordo semplicemente a tutti voi, la maggior parte dei quali miei coetanei,

In conclusione, quello giunto dal Governo era un testo con poche luci e tante ombre che il proficuo lavoro del Senato, un lavoro serio, costruttivo, nel merito e meticoloso è riuscito a rendere più luminoso. Annuncio dunque, nonostante persistano ancora zone d'ombra, ma ritenendo

la valutazione che il Gruppo Articolo 1- Movimento Democratico e Progressista esprimerà nei confronti del decreto che oggi votiamo poggia su due premesse fondamentali. prima: siamo favorevoli ai vaccini. Li consideriamo, come già ricordato dalla senatrice Dirindin nel suo intervento, uno strumento indispensabile di prevenzione delle malattie infettive e di contenimento della morbilità e della mortalità. seconda: non pensiamo che la vaccinazione possa essere sempre e esclusivamente affidata alla libera scelta dei cittadini. Nel campo delle malattie trasmissibili le scelte dei singoli hanno infatti conseguenze sulla collettività che devono essere tenute in considerazione e possono rendere necessario il ricorso a misure di coercizione della libertà individuale come sono gli obblighi vaccinali. Lo strumento dell'obbligo non deve, però, mai essere considerato come il solo strumento da adottare, neppure quando lo si consideri necessario in ragione di un alto rischio di contagio. Per questo motivo abbiamo condiviso,

Per questo motivo abbiamo condiviso e ancora condividiamo l'impostazione indicata nel Piano nazionale

Ristabiliamo la tranquillità dell'Aula. Questo è un dibattito serio, un dibattito difficile. Cerchiamo di essere rispettosi l'uno con l'altro e di dimostrare la nostra serietà. Colleghi, è responsabilità di tutti. Vorrei che la senatrice Guerra potesse continuare il suo intervento. *(Commenti Senatore D'Anna, questo è l'ultimo richiamo. Altrimenti, dovrò pregarla di lasciare l'Aula. La prego di stare tranquillo. Andiamo avanti.

la valutazione che il Gruppo Articolo 1- Movimento Democratico e Progressista esprimerà nei confronti del decreto che oggi votiamo poggia su due premesse fondamentali. La prima: siamo favorevoli ai vaccini. Li consideriamo, come già ricordato dalla senatrice Dirindin nel suo intervento, uno strumento indispensabile di prevenzione delle malattie infettive e di contenimento della morbilità e della mortalità. seconda: non pensiamo che la vaccinazione possa essere sempre e esclusivamente affidata alla libera scelta dei cittadini. Nel campo delle malattie trasmissibili le scelte dei singoli hanno infatti conseguenze sulla collettività che devono essere tenute in considerazione e possono rendere necessario il ricorso a misure di coercizione della libertà individuale come sono gli obblighi vaccinali. Lo strumento dell'obbligo non deve, però, mai essere considerato come il solo strumento da adottare, neppure quando lo si consideri necessario in ragione di un alto rischio di contagio. Per questo motivo abbiamo condiviso, e ancora condividiamo, l'impostazione indicata nel Piano nazionale.

Siamo pronti a ristabilire l'ordine? Prego

Lo strumento dell'obbligo non deve, però, mai essere considerato come il solo strumento da adottare, neppure quando lo si consideri necessario in ragione di un alto rischio di contagio. Per questo motivo abbiamo condiviso e ancora condividiamo l'impostazione indicata nel Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019, approvato solo qualche mese fa. Una impostazione fondata sull'idea di accompagnare i cittadini, attraverso l'educazione sanitaria, l'informazione e la responsabilizzazione, a un'adesione il più possibile volontaria e comunque sempre consapevole, piuttosto che sull'esercizio di un potere coercitivo. Purtroppo, il decreto-legge che oggi ci apprestiamo a convertire non si è posto in continuità con questo approccio. La scelta più critica e discutibile è stata quella di estendere in modo drastico l'obbligo vaccinale, accompagnando tale scelta con la previsione di una struttura sanzionatoria che è apparsa subito eccessiva. La scelta compiuta è stata motivata con riferimento al calo registrato nelle coperture vaccinali che (sicuramente per il morbillo) ha portato al di sotto delle soglie considerate necessarie per non compromettere l'immunità di gregge. Non altrettanto dirimente è risultata l'evidenza messa a disposizione del Parlamento per quanto riguarda le altre sette vaccinazioni rese obbligatorie, ridotte poi a cinque, e affiancate dalla giusta previsione di un successivo monitoraggio. L'impostazione seguita conteneva poi incoerenze, in parte sanate nel percorso parlamentare, come la mancata estensione dei nuovi obblighi vaccinali a persone, quali gli operatori sanitari e della scuola, che possono contribuire alla trasmissione del contagio. Il percorso parlamentare è stato importante anche nell'introdurre altre modifiche, a cui hanno concorso più Gruppi parlamentari tra cui, attraverso il lavoro tenace, puntuale e competente della senatrice Dirindin (che ringrazio), anche il nostro: modifiche che hanno indubbiamente concorso a determinare

anche perché il bilancio fra i costi sociali e personali che può imporre e l'efficacia che ne può scaturire pende drammaticamente a favore dei primi. Ricordo in secondo luogo un insieme di previsioni che hanno rafforzato e migliorato il piano di attuazione delle norme introdotte: e il coordinamento fra ASL e scuole nella predisposizione e trasmissione delle certificazioni, dall'altro, che abbiamo fortemente voluto e che dovrebbe, in prospettiva, ridurre i costi di adempimento posti in capo ai cittadini. Questi costi sono stati in parte attenuati anche con l'introduzione di norme transitorie. Esprimiamo invece insoddisfazione per il compromesso raggiunto sui vaccini monocomponenti, cui si potrà fare ricorso solo «di norma» e «nei limiti della disponibilità del servizio» e che rischia quindi di tradursi in un mero palliativo. Giudichiamo positive, per quanto ancora timide, le aperture introdotte relativamente alla farmacovigilanza. Si è trattato nel complesso di emendamenti importanti, per quanto costruiti al di fuori di un quadro organico, quel quadro che mancava alla stesura originaria del decreto-legge. Per questo, nel processo di attuazione della norma, la nostra vigilanza e il nostro monitoraggio saranno costanti. È nostra convinzione, infatti, che la riduzione dei costi di adempimento giochi un ruolo importante nel favorire quell'adesione volontaria ai vaccini che consideriamo, come detto, prioritaria. Altre considerazioni critiche merita la conduzione dell'*iter* parlamentare: si è scelto di privilegiare un accordo politico al di fuori della maggioranza, con Forza Italia, da cui siamo stati esclusi, pur essendo noi una competente della maggioranza. un accordo che ha avuto, a più riprese, il sapore dello scambio piuttosto che quello della giusta ricerca di un allargamento del consenso: ne è testimonianza, ad esempio, l'accanimento con cui si è cercato, attraverso la predisposizione di formulazioni sempre nuove, tutte bocciate dalla Commissione bilancio in quanto qualche regalo alle farmacie, addirittura ipotizzando la somministrazione dei vaccini all'interno delle stesse. Non è stato dato alcun chiarimento in merito al potenziale conflitto di interessi, che è stato oggetto di una nostra interrogazione urgente e che è stato ricordato e illustrato nel suo intervento dalla senatrice Dirindin. In conclusione, nell'esprimere il voto a favore del decreto-legge da parte del Gruppo Articolo 1 - MPD, devo sottolineare che gli elementi critici a cui ho fatto riferimento e, in particolare, le preoccupazioni sollevate in alcuni membri del Gruppo dalla scelta *core* del provvedimento, di portare da quattro a dieci il numero dei vaccini obbligatori, non hanno permesso di giungere ad una piena omogeneità di vedute. Si tratta di temi che coinvolgono non solo valutazioni tecniche e scientifiche, ma anche convincimenti profondi e soggettivi, che il Gruppo Articolo 1 - MDP intende rispettare, dando quindi pieno riconoscimento all'espressione di voti in dissenso.

Signora Presidente, signora Ministro, colleghe e colleghi, avrei desiderato che questo confronto si svolgesse in un clima differente, mentre il dibattito, le dichiarazioni e le valutazioni sono stati accompagnati dall'eco sgradevole di atteggiamenti e finanche da provocazioni che, come abbiamo visto poco fa, offrono uno spettacolo non edificante del nostro ruolo.

senza pregiudizio, ma non senza preoccupazioni o incertezze. Lo dico molto chiaramente: lo abbiamo siamo favorevoli ai dubbi generatori di verità, ma siamo fortemente contrari, soprattutto quando... *(Brusio).* Chiederei cortesemente ai colleghi che sono alla mia sinistra di consentire lo svolgimento del mio intervento.

alle contese politiche che si alimentano di insinuazioni, che veicolano disinformazione e generano confusione e sgomento. Vedete colleghi, qualche giorno fa una mamma, che ha parlato rompendo il silenzio di quella enorme platea, maggioritaria nel Paese mi permetto di dire, che sostiene con responsabilità la cultura vaccinale, ha scritto una lettera al Presidente Grasso e ha chiesto una cosa molto semplice (peccato che sia stata chiesta, perché dovrebbe essere insita nelle abitudini di questa ha detto che un legislatore deve essere dotato di qualità morali che non devono vacillare al primo sussulto di piazza; di aver ascoltato tra gli scranni del Senato parole che fanno tremare i polsi e rivelano quanto radicate siano l'ignoranza e la scaramanzia. Sono parole severe, Sono parole severe, che interrogano le nostre coscienze e devono spingerci a capire che, forse, abbiamo ancora la possibilità di riconciliare la piazza al Palazzo se noi qui, oggi, in quest'Aula, recuperiamo il valore e il senso di una funzione al servizio del Paese e facciamo in modo che il dibattito maturo e responsabile che in quest'Assemblea si realizza sia lo strumento attraverso il quale raggiungere un obiettivo, al di là delle posizioni differenti, facendo avvertire al Paese non la contesa, ma lo sforzo di raggiungere un obiettivo comune su un tema che riguarda la salute dei cittadini italiani. italiani. Questo è l'atteggiamento che noi abbiamo avuto. Certo, signora Ministro, come ho ripetuto più volte in altri interventi e in Commissione, sarebbe stato preferibile un disegno di legge al posto di un decreto-legge, che ha un effetto imperativo e detta tempi particolarmente

coerente declinazione di una maggiore responsabilità sul piano dell'informazione, dell'educazione e della divulgazione di principi scientifici ai quali noi ci siamo attenuti nel dibattito e nella costruzione degli emendamenti correttivi. Abbiamo ragionato senza pregiudizi, perché la scienza non è un *optional*. Siamo convinti che la buona politica - perché esiste la buona politica - accompagni la scienza, accompagni le decisioni che devono essere alimentate e supportate dalla ricerca ricerca scientifica e da quello che le autorità preposte diffondono a livello internazionale e ci dicono che la vaccinazione e la potabilizzazione dell'acqua sono le due più straordinarie conquiste che abbiamo potuto fare negli ultimi secoli. Così come la migliore misura di prevenzione per la tutela della salute resta quella vaccinale. C'erano dei punti di criticità, ma devo dire che con un dibattito faticoso e un confronto, talvolta anche aspro, si sono fatti alcuni passi in avanti. alla cessazione dell'obbligo dopo tre anni, all'attivazione di un'attività di monitoraggio, valutazione e diffusione degli eventi avversi. Tutto ciò al fine di sgombrare il campo, perché non è possibile pensare che si voglia nascondere qualcosa a qualcuno: questo è offensivo solo a pensarlo.

le misure orientate allo sviluppo di un'attività d'informazione, di educazione e di formazione, che sono presupposti irrinunciabili perché generano la consapevolezza, la scelta matura, consapevole, libera e responsabile della nostra comunità. Infine, cito la copertura vaccinale per i minori stranieri, l'anagrafe nazionale per un attento monitoraggio

sia stato già chiarito come e quanto taluni interventi siano fortemente ancorati a un'inimicizia nei riguardi di chi sottoscrive emendamenti a sostegno del ruolo sociosanitario e assistenziale della farmacia. Ognuno farà i conti con la propria coscienza e con il proprio modo di legiferare. Siamo convinti che la politica, per essere una buona politica, debba declinare necessariamente il principio di responsabilità. prioritario ci siamo rifatti nella consapevolezza che la responsabilità politica, al di là delle differenti posizioni che confermiamo di contrarietà rispetto al Governo in termini generali, ci fa riconoscere nella vaccinazione un atto intimamente connesso ai principi di universalità e solidarietà, perché la vaccinazione del singolo non è soltanto mezzo di tutela della salute dello stesso, ma diventa un imprescindibile modo di copertura e di garanzia per l'intera comunità.

in tutte le possibilità che avrà di distillare nel Paese una cultura di consapevolezza. Si passi dalla cultura dell'obbligo alla cultura dell'adesione consapevole. Per farlo dobbiamo fare una crociata di informazione tanto più grande e imponente quanto maggiore è stata la voce che si è levata nelle piazze da parte di ciarlatani, figli di una teoria teoria assolutamente oscurantista e medievale che noi contrastiamo fermamente. Per queste motivazioni esprimo il prudente voto favorevole della componente dei senatori di Direzione Italia.

il lungo e articolato dibattito in Commissione sanità e in Aula mi limiterò a riprendere due aspetti principali contenuti in questo decreto vaccini, che di fatto ne caratterizzano la valenza sia scientifica che politica: la necessità di ripristinare l'obbligo vaccinale e l'ampliamento delle vaccinazioni obbligatorie. I due profili sono strettamente collegati tra loro e conseguenti ai dati epidemiologici che ci sono stati comunicati, sostanzialmente a una ripresa preoccupante di alcune malattie infettive per la salute pubblica nel nostro Paese e nel mondo e la riduzione purtroppo in Italia in pochi anni delle coperture vaccinali. Durante il dibattito ho sentito diversi interventi anche di colleghi medici - io sono medico di medicina generale - che considerano poco significativi, inattendibili e quasi banali i dati e lo stesso operato dell'Istituto superiore di sanità. Ritengo che questo atteggiamento sia poco comprensibile. Perché contestare solo i dati scientifici epidemiologici sui vaccini e non dire assolutamente nulla sui protocolli e sui documenti scientifici sulle malattie metaboliche, oncologiche o di prevenzione?

riguardo alle epidemie che colpiscono i bambini nel mondo e alla necessità di rinvigorire le campagne vaccinali. Ricordo altresì l'atteggiamento positivo dell'Organizzazione mondiale della sanità verso il provvedimento in Tornando al decreto-legge, credo ci siano buone ragioni per alzare la guardia sui vaccini, come dimostrato dagli studi cui ho accennato. Praticamente tutte le vaccinazioni sono sotto la soglia dell'immunità di gregge del 95 per cento e, come è già stato detto, le coperture vaccinali italiane sono tra le più basse d'Europa: non mi sembra poco. poco. La reintroduzione dell'obbligo vaccinale - e mi viene da pensare che forse nel 1999 sarebbe stato meglio non eliminarlo - ha quindi lo scopo di porre all'attenzione dei cittadini una criticità che interessa la salute pubblica, che coinvolge sia i più piccoli

Analogamente, anche rispetto all'ampliamento delle vaccinazioni obbligatorie, oggetto oltretutto di non fondata preoccupazione dei cittadini, rilevo che da anni proprio grazie ai piani vaccinali nazionali i bambini ricevono 9-10 vaccinazioni e non è successo nulla da decenni. Questo lo considero un atto concreto volto alla riduzione costante delle più comuni malattie infettive e delle loro complicanze più insidiose, con benefici indiretti per le fasce di popolazione in cui sono rappresentati sempre di più gli ammalati cronici, i diabetici, i cardiopatici, i pazienti oncologici, cioè persone che non potranno che beneficiare di questo risultato.

la possibilità di vaccinazioni monocomponenti, per le quali personalmente nutro qualche dubbio; l'eliminazione della previsione di sospendere la patria potestà in caso di resistenza alla norma. Sottolineo inoltre l'accoglimento dell'emendamento della senatrice Cattaneo riguardo a precisazioni e modifiche degli aspetti

necessario per il bene e la tutela della salute pubblica. Ribadiamo l'assoluta validità delle vaccinazioni e il loro formidabile ruolo storico come indispensabile atto medico per le più insidiose malattie infettive e per la salvaguardia della salute di milioni di persone, anche alla luce dei recenti e grandi movimenti migratori. Come senatori delle autonomie speciali diamo grande importanza

Statuti speciali non sono inseriti nella Costituzione italiana. Poniamo inoltre grande importanza nelle azioni di farmacovigilanza rinforzate dal decreto-legge, per tutelare al massimo la popolazione verso possibili effetti avversi. Ricordo che non esiste in medicina e in chirurgia alcun intervento che abbia pericolo di complicanze uguale a zero. Quindi, con il cuore leggero, confortato dalla memoria di scienziati come Louis Pasteur e Albert Sabin e proprio con lo spirito del grande scopritore del vaccino contro la poliomielite, che decise di regalare il suo brevetto

è accompagnato dal sindaco di Isola del Liri, che è gemellato con il comune di New Orleans. Buongiorno sindaco. Ringrazio la senatrice Spilabotte, che ha fatto incontrare questa delegazione con la Presidenza.

Ad esempio, se qualcuno la pensa diversamente rispetto a un altro senatore, è soggetto a ingiurie e a epiteti inaccettabili. Questo veramente, per quanto ci riguarda, è una cosa assurda e inconcepibile. Noi crediamo che durante il dibattito molte volte ci sia stata arte.

Lo diciamo, per quanto ci riguarda, non senza sentire il dovere di precisare che paradossalmente sono emerse tesi strane, in un clima strano: tesi che prevalgono sulle prove scientifiche, sul buon senso, sulla necessità di garantire la salute collettiva. Sono emersi chiari ed evidenti elementi di strumentalizzazione, di mera strumentalizzazione. Noi rimaniamo convinti ancor di più, anche sulla base di meline estenuanti, che a valere siano solo e soltanto le valutazioni scientifiche e istituzionali, le quali confermano che attualmente nei vaccini in commercio, ad esempio, già dal 2002 non ci sono più derivati del mercurio. Inoltre, confermano fortemente che le quantità di formaldeide e di alluminio tanto sbandierate sono solamente minimali, da non causare assolutamente alcun danno alla salute. E, ancor di più, esse sono di molto inferiori in concentrazione anche rispetto a ciò che quotidianamente mangiamo ovvero beviamo con le più note acque oligominerali in commercio. Non esiste una sola prova di laboratorio che certifichi e che dimostri la presenza di metalli pesanti in quantità anche lontanamente tossiche, tanto meno per quanto riguarda il tungsteno,

sono emersi dei dati inequivocabili, cioè: nessun caso. Non fomentiamo, non diamo notizie errate, non creiamo sgomento senza avere conoscenza di basi scientifiche. La sicurezza dei vaccini è documentata da milioni di dosi somministrate, dalla costante attività di sorveglianza delle agenzie regolatorie ed anche dell'industria, prima dell'immissione in commercio. Vorrei qui fare un piccolo esempio, signora

altri, circa due miliardi di euro per sostanze omeopatiche e poi rifiutiamo dei vaccini innocui, con una disinformazione veramente artata. Il risultato di cotanta disinformazione è che ad oggi ci troviamo, guarda caso, con i reparti di malattie infettive pieni, non c'è più un posto letto libero. Le conseguenze di

riguarda soggetti non vaccinati, il 6 per cento addirittura soggetti che hanno avuto una sola dose di vaccino. Nel 41 per cento dei casi è stato necessario il ricovero, con le conseguenze prima citate.

Si fa riferimento ad una scheda, nel caso di specie, inserita nel 2009 come trattamento per terapia anticonvulsivante. Sei mesi dopo la scheda veniva aggiornata con il decesso,

come prova provata, c'è da precisare che il sito della Food and Drug Administration riporta il ritiro di un solo lotto a scopo meramente precauzionale per un problema squisitamente meccanico nella fase di riempimento asettico. tratta quindi di un problema sorto nella fase di preparazione. Questo lotto non risulta distribuito in Italia ed anche un altro lotto che era indirizzato alla Francia è stato ritirato sempre per difetti meccanici.

Cito un'ulteriore inesattezza, signora Ministro, anche per sgomberare il campo dalle solite strumentalizzazioni: c'è chi accusa Aifa di non fornire i dati

che Aifa fornisce tutti i dati perché il suo primo interesse è la tutela della salute collettiva. Il numero delle reazioni avverse segnalate nel rapporto rappresenta un insieme di tutto quanto è avvenuto in Italia; i dati sono elaborati su basi scientifiche e non ammettono errori. Il numero delle reazioni avverse va letto in modo oggettivo, e cioè: i vaccini, considerati farmaci biologici, così come qualsiasi altro farmaco possono produrre effetti indesiderati; nel caso dei vaccini vengono registrati puntualmente

I dati raccolti accuratamente testimoniano la correttezza procedurale nonché l'assoluta sicurezza dei vaccini. Ci sono anche altre cose aberranti. Abbiamo sentito parlare in quest'Aula di stimolazioni immunitarie anomale, atipiche, di presenza di estratti umani: veramente assurdo. Quale supporto scientifico esiste nel merito? Io credo che ci si dovrebbe vergognare a fare questo tipo di considerazioni! SANGALLI *(PD)*. Bravo. L'ufficio per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità è preoccupato per la situazione difficile che si è creata in Italia, con la diffusione soprattutto del morbillo in modo quasi ingravescente e anche di altre malattie prevenibili con i vaccini, di cui non si è parlato. Nessuno parla, ad esempio, di ricoveri di osteomieliti o di encefaliti conseguenti a patologia morbillare. Il tasso di immunizzazione è sceso vertiginosamente. Questo decreto, invece, non è passato inosservato a livello internazionale, tant'è vero che il direttore generale dell'OMS regionale ha espresso plauso

Soffermiamoci sulle principali modifiche introdotte in sede di conversione. In questo caso possiamo sì parlare di un dibattito costruttivo. Quanto alle modifiche introdotte - innanzitutto mi riferisco alla rimodulazione degli obblighi vaccinali la discussione qui è stata seria e costruttiva ed ha consentito di migliorare il testo *(Commenti dal Gruppo M5S )* stabilendo che una rimodulazione degli obblighi vaccinali possa risultare più aderente alla complessa situazione epidemiologica del Paese e, nel contempo, più sostenibile da parte delle famiglie.

Da qui dunque la scelta di considerare obbligatorio il vaccino tetravalente, senza escludere che in futuro detto obbligo possa venire meno,

abbiamo ascoltato l'imbarazzante intervento della ministra Lorenzin. Nella guerra tra populismi sui vaccini, lei è lì a combattere per una parte. Ora è chiaro perché è stato deciso di prevaricare ancora una volta il ruolo del Parlamento, privandolo della potestà legislativa ordinaria e imponendo un decreto-legge: una piena violazione della Costituzione, del diritto alla salute, della libertà di scelta consapevole e quello all'istruzione; un vero disastro culturale e sociale,

quindi risparmiamoci la retorica del voi non sapete quante malattie sono state sconfitte o i racconti di tragedie umane che purtroppo conosciamo direttamente tutti noi. I vaccini sono importanti interventi di salute pubblica, fondamentali per sconfiggere la morbilità e la mortalità di alcune malattie infettive e un mezzo efficace di prevenzione. Dover fare questa premessa la dice lunga sul clima di intolleranza, caccia alle streghe che si è sviluppato nel nostro Paese, una discussione da curva da stadio (a partire dalle argomentazioni della Ministra) e solo pochi, molto pochi, si sono soffermati sul merito del decreto. La nostra discussione non può essere banalizzata tra chi è contro i vaccini e chi è a favore. La discussione in quest'Aula, se fosse stata ascoltata anche dalla Ministra, è stata seria e si è avuto un confronto utile, come dimostrano i seppur pochi emendamenti approvati. Non sarà certo un decreto-legge del Governo a far cambiare improvvisamente opinione a chi nutre dubbi, scetticismo e ha scelto di non vaccinare o fare solo alcuni vaccini ai propri figli. Ma la propaganda di Stato ha scelto questa modalità comunicativa per distogliere l'attenzione da un decreto fatto male, espressione della peggior tecnocrazia sanitaria e mette in evidenza la pessima condizione di un servizio sanitario pubblico (servizi vaccinali compresi) che non è in grado prendere in carico la salute dei cittadini, ma soprattutto di far crescere la consapevolezza del bisogno di salute. Questo è il cuore della discussione. Noi non ci faremo trascinare in alcuna crociata: quelle le lasciamo alla Ministra e a chi, nella maggioranza, ha scelto quella guerra. Se i vaccini sono importanti, perfettibili ma irrinunciabili, allora allora perché la responsabile del dicastero della Salute non ha pensato ad una grande campagna di comunicazione, informazione e formazione rivolta ai cittadini, agli operatori sanitari del servizio sanitario pubblico, piuttosto che irridere i cittadini? Comprendiamo che dopo ben due tentativi falliti di campagne sul Fertility Day avrebbe avuto qualche difficoltà, ma sarebbe stata più utile la presa in carico anche della cultura sanitaria dei propri cittadini. Secondo il Ministero siamo dinanzi ad un calo delle coperture vaccinali, ma non si dichiara alcuna emergenza. D'altra parte lo stesso *premier* Gentiloni Silveri ha detto che non esiste emergenza. Eppure le coperture vaccinali erano in diminuzione da un po' di tempo, ma non è stato dato alcun allarme, forse perché siamo nel calo fisiologico? I tanti esperti incontrati e ascoltati hanno confermato che non esiste un'emergenza nazionale. Nel 2011 (anche quel Governo era sempre sostenuto dal partito della Ministra) fu registrato lo stesso calo sul morbillo, ma il fatto non creò alcuno scossone nella politica. Dunque, cosa è accaduto? Perché dal 2003, quando è stato messo in atto il piano contro il morbillo, i dati non sono migliorati ma nemmeno peggiorati? Perché se l'età media è ventisette anni non abbiamo messo in atto un piano vaccinale soprattutto per gli adulti? La Ministra ha parlato di migliaia di morti per il morbillo. Vorremmo conoscere la fonte di quei dati. De Pin e Simeoni)*. I pediatri del servizio sanitario nazionale hanno raccontato che lo scetticismo e la diffidenza nei confronti dei vaccini esiste da sempre, ancora prima della nascita dei no vax, dei *free* vax e non solo in Italia. I pediatri, però, hanno raccontato il profondo senso di solitudine perché il servizio sanitario nazionale pubblico li ha lasciati soli a prendersi cura della responsabilità genitoriale oltre che della salute dei cittadini. Non sono riusciti - ma era impossibile riuscire - a frenare quella frattura tra cittadini e scienza, tra cittadini e Servizio sanitario nazionale. Perché la Ministra non ha cercato di capirne le cause avvalendosi delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale sanità? Dove e quando si è rotto il rapporto di fiducia tra cittadini e scienza, tra cittadini e Servizio sanitario pubblico? Perché i cittadini non si sentono protetti e accolti dal Servizio sanitario nazionale? Cosa si è rotto nel rapporto tra Servizio sanitario nazionale e medici di famiglia? Perché non siamo stati trasparenti ed evitato di nascondere gli eventi avversi dei vaccini distinguendo tra rischi e probabilità? Perché abbiamo obbligato i piccoli a dosi eccessivi multiple senza dare la possibilità e la libertà di scelta di tempi e modi diversi? Aver previsto dosi monocomponenti per gli immunizzati è stato sicuramente un piccolo passo avanti, ma perché non prevederlo per tutti i vaccini? Sono aspetti importanti e utili a rassicurare. Sopratutto, perché non si è scelto di fare una campagna contro la corruzione, gli intrecci tra multinazionali del farmaco e sanità? Questo, negli ultimi anni, ha avuto un ruolo *(Applausi della senatrice Simeoni)*. Una Ministra attenta alle politiche della famiglia avrebbe dovuto sapere che qui parliamo di responsabilità genitoriale che non può essere delegata. Lo Stato, a meno che non dichiari lo stato di emergenza, non può sostituirsi, ma si tratta di far crescere cultura e consapevolezza del bisogno di salute e cultura della salute. Certo, tutto più faticoso, ma unica strada se vogliamo far crescere cittadini sovrani e non cittadini sudditi, come sosteneva il così tanto citato in questi giorni don Milani. Ma non mi sembra la strada scelta da una Ministra che alimenta lo scontro e considera i dubbiosi e gli scettici nemici, non cittadini di cui farsi carico. Vorremmo chiedere alla Ministra come è stato pensato di rendere efficiente il Servizio sanitario nazionale, laddove necessario per assolvere all'obbligo vaccinale. Immagino siano state previste risorse per assunzioni (non ingaggi, Ministra) di infermieri, medici, personale sanitario, risorse per la riapertura dei presidi territoriali, dei consultori che in molte zone del nostro Paese sono stati chiusi o svuotati di funzioni perché avete fatto tagli tremendi alla sanità. Dove sono le risorse a copertura dei vaccini? Aver scritto gratuiti nel testo di legge non vuol dire che non sono e non saranno previsti *ticket*. E con quali risorse si pagheranno gli esami del sangue per trovare i segni dell'avvenuta immunizzazione? Se queste cose non ci sono, parliamo del nulla. E per fortuna è stato scongiurato il salto in farmacia per un vaccino. Certo, è l'unico ordine del giorno approvato in questi quattro anni che non parla di «valutare l'opportunità».

Il decreto-legge specifica che l'attuazione spetta alle Regioni, che in virtù della propria autonoma organizzazione sanitaria sceglieranno se dare seguito al decreto-legge. Persino l'erogazione e la riscossione della sanzione spettano alle Regioni e siamo curiosi di capire cosa accadrà in quelle Regioni che hanno escluso l'uso di sanzioni, o cosa accadrà in Trentino-Alto Adige, dove si invoca l'autonomia statutaria - giustamente - per sottrarsi a questo decreto-legge. Peccato che i loro rappresentanti votano per la nostra obbligatorietà.

che non hanno fatto vaccini e che magari saranno in coda alle ASL in attesa di farli. Non è un caso che la ministra Fedeli si sia affrettata a dire «abbiamo annunciato», senza spiegare nel giro di quarantotto ore, mettendo in dubbio il diritto costituzionale al diritto allo studio. Negate l'accesso alla scuola dell'infanzia? Gravissimo. Questa sarebbe la vostra buon scuola? Ci saremmo aspettati una sollevazione da parte del mondo della scuola, degli insegnanti, dal personale ATA e dai dirigenti scolastici, ai quali spetterà il compito di controllare la regolarità vaccinale e soprattutto di presentare le proprie certificazioni vaccinali, altrimenti analisi a pagamento. Naturalmente, se si vive nelle Province di Trento e Bolzano, lì si fa solo una promozione sulle adesioni vaccinali. Per non parlare della sanzione pecuniaria che, per quanto ridotta, è il segno evidente che pensate a una società classista, dove chi ha, può tutto, e chi non ha deve subire. L'approccio coercitivo è tipico di Paesi arretrati, in perfetta linea con la scelta di verticalizzazione autoritaria che abbiamo visto esplicarsi nella vostra proposta di riforma costituzionale. Ma forse avete dimenticato velocemente che quella riforma è stata bocciata dai cittadini. Resterà un mistero perché il Partito Democratico abbia deciso di subire questo decreto, voluto da una Ministra di altro partito. Le uniche modifiche apportate sono in virtù dell'accordo con Forza Italia che rivendicherà i miglioramenti. Al Partito Democratico resterà la responsabilità di questo pasticcio. Prendo in prestito le parole di un ricercatore dell'istituto Mario Negri che, commentando il decreto, ha detto: «C'è una grande differenza fra l'obbedienza cieca alle regole e l'obbedienza illuminata dello spirito critico». Noi scegliamo quest'ultima. Noi non siamo contro i vaccini, ma voteremo contro questo decreto, che conferma soltanto che il Ministero della salute è senza

Signora Presidente, colleghi, sono più di quattro anni che è cominciata la nostra esperienza in Parlamento e ne abbiamo viste tante. Gli addetti ai lavori, funzionari, assistenti, dicono che una legislatura come questa non ha avuto precedenti. Volevate trasformarla in una Costituente: proprio voi, siete la coda di decenni di abusi di potere ai danni del popolo italiano, fino a quello di non mandarci a votare, tra maggioranze ricostruite e ristrutturate, al solo scopo di non schiodare da una poltrona. Ma non eravate contenti. Dopo aver inanellato una serie interminabile di fallimenti (e ne ricordo alcuni: il *jobs act*, la buona scuola, la legge elettorale, miliardi e miliardi per salvare le banche, la truffa ai correntisti), non contenti, volevate concludere, come si dice a Roma, con il botto. E così avete fatto un bel decreto-legge sull'obbligo vaccinale, che con il clima che c'è nel Paese ha sortito l'effetto, quasi ovvio, di un *boomerang* che pagheremo tutti a caro prezzo. Vede, infatti, signor Ministro...

Vede, Ministro, mentre lei andava in televisione, parlando di *virus* che infettano ed uccidono, sparando numeri a caso, attribuendo epidemie in luoghi sparsi del globo e mettendoci in guardia sul tetano, se cala l'immunità di gregge, tanti genitori, tanti italiani che spesso sono distratti, stanchi dei discorsi vuoti di questa politica, hanno drizzato le orecchie. Agli italiani puoi toccare tutto, ma continuano ad avere verso i propri figli quell'immenso senso di protezione che ha reso le madri italiane famose nel mondo, quelle che sanno se il figlio non si sente bene da come piega la testa o solo guardandolo negli occhi. Quelle mamme oggi sono insegnanti, dottoresse, laureate e stimate professioniste, che probabilmente hanno avuto il loro bambino ormai quarantenni perché prima non potevano, visto che questo Stato non ha fatto nulla per poter far garantire loro un mondo degno ai propri figli. figli. Queste mamme, Ministro, questi genitori, che si informano, che leggono, che si pongono delle domande, quelli che ho sentito definire vaccinoscettici (forse per un eccessivo senso di protezione nei confronti dei propri figli, quel senso di protezione che voi avete etichettato come ignoranza, credulità, dabbenaggine), quei genitori si sono fatti delle domande. E lei, Ministro, a quelle domande ha risposto con la delicatezza di un *panzer*, annunciando *urbi et orbi* che, a causa di una epidemia di morbillo, sarebbero stati introdotti dodici vaccini obbligatori e che i bambini non vaccinati non sarebbero stati ammessi ai nidi e alle materne. Inizialmente, lei voleva togliere loro anche il diritto all'istruzione, ma poi la sua collega Fedeli, sedutale ora accanto, le ha fatto presente che stava leggermente esagerando! avete optato per la sanzione ai genitori. Ma non una sanzione da poco: 7.500 euro, e se non vaccini, ti levo pure il figlio. Voi siete dei pazzi. E cosa vi aspettavate che sarebbe accaduto? Vi siete presentati con un decreto-legge così folle e impresentabile che quest'Assemblea, signor Ministro, glielo ha smontato pezzo per pezzo, certificando - semmai ce ne fosse ancora bisogno - il suo totale fallimento politico come Ministro della salute. Ce li ricordiamo bene i suoi atti da Ministro in questi cinque anni: ha dedicato la sua attività a nobili cause, come il taglio di 4 miliardi al Servizio sanitario nazionale, ha dimezzato le prestazioni in convenzione con il disegno di legge appropriatezza e anche in quel caso - è un po' un suo vizio - aveva cominciato minacciando multe ai medici che avessero prescritto analisi o esami diversi da quelli che lei aveva deciso che servissero; poi si è dedicata al Fertility day e quello dovevamo coglierlo come un segnale, perché per lei la donna è un'ovaia a forma di clessidra che va a tempo e l'uomo è uno spermatozoo sempre attivo fino agli ottant'anni. Insomma, lei, Ministro, che in questi cinque anni avrebbe dovuto gestire quella che sta presentando oggi come un caposaldo della tutela della salute, ci viene a raccontare che nel Paese c'è un'epidemia di morbillo

che si richiedeva la vaccinazione per il morbillo al fine di tutelare la salute pubblica. Le dico di più: poteva dire che sarebbe stata somministrata prioritariamente a tutti i bambini, da zero a

tutti coloro che appartengono al comparto della scuola e al comparto sanitario, cosa per la quale invece ci avete detto che non c'erano i soldi. Vaccinate i nostri figli perché potete ricattare i genitori e non vaccinate invece coloro dai quali vi aspettate un voto: siete sempre forti con i deboli, ma estremamente deboli con i forti. Ecco, Ministro, un Paese si aspetta che un Governo serio faccia questo, quando c'è un'epidemia in atto che può provocare la morte. Ma voi non lo avete fatto. veramente accadesse una cosa del genere non potreste neanche operare, come le ho detto, perché siete in grado di imporre dieci vaccini, ma non siete in grado di garantirne uno solo. In quest'Aula ci è stato risposto

Ministro, le dico anche che forse la pericolosità di alcune patologie non è più percepita come tale, perché sono state debellate e anche grazie ai vaccini. Ma piuttosto che addossare la colpa ai genitori, che secondo questo Stato dovrebbero essere medici, giuristi e commercialisti, perché tanto dobbiamo fare tutto da soli, lei, Ministro, avrebbe dovuto operare affinché questa consapevolezza divenisse tale. E avrebbe dovuto farlo informando, aprendo un dialogo. Ministro, tolga da questo decreto ogni coercizione e multa. L'attenzione sul problema del calo delle coperture vaccinali è stata, anche se in modo maldestro, attirata. Teniamo in piedi tutto quello che concerne l'Anagrafe vaccinale, la farmacovigilanza, ma anche la collaborazione con la scuola per raccogliere più velocemente i dati, considerando che solo oggi, nel 2017, si parla di un'Anagrafe nazionale, in maniera tale da garantire che, anche nelle classi dove vi siano soggetti fragili, vi sia la giusta garanzia di tutela. Chiamiamo i genitori che per motivi a voi ignoti hanno ritardato o omesso una vaccinazione; parliamo con loro, capiamo le loro ragioni e offriamo ai nostri figli il rispetto che meritano. Scegliamo di accompagnare questi genitori verso la vaccinazione in modo che diventi una scelta consapevole, un atto volontario.

tabella sono Paesi europei, dove non è prevista l'obbligatorietà, ma è prevista la raccomandazione e le loro coperture vaccinali sono migliori delle nostre. *(Applausi Vuole sapere perché gli altri Governi possono permettersi di non imporre le vaccinazioni, ma di raccomandarle e, in questo modo, raggiungere una percentuale di vaccinazioni tanto alta? Perché i loro cittadini si fidano delle istituzioni. In Italia non è così. I genitori sono ormai disorientati dalle loro domande senza risposte, da un obbligo, una multa o dalla possibile perdita dei figli; insomma, questi genitori, non avendo risposte hanno cominciato a cercarle sui giornali, hanno seguito i lavori d'Aula e lo sa che cosa hanno visto? Hanno visto una trattativa sul numero dei vaccini che erano importanti o no: da dodici a dieci e non si è mai capito il perché. L'obbligo per il meningococco non esiste in alcun Paese europeo, ma forse erano queste le politiche industriali che interessavano al Governo italiano, non certo quelle della tutela della salute dei nostri figli. E comunque hanno visto la trattativa marchetta per le farmacie, nonché la marchetta per le scuole, insomma la trattativa sulla pelle dei loro figli. Ministro, voci più autorevoli della mia hanno evidenziato in Commissione dubbi su tempi e modi di questo decreto. Hanno sollevato dubbi sulla reale necessità di alcune delle vaccinazioni che lei sta rendendo obbligatorie. Lei si sta assumendo la responsabilità che è di ogni genitore, ossia quella di volere il meglio per il proprio figlio. Ministro, glielo dico sinceramente: non credo che lei abbia pienamente compreso la gravità della sua azione, ma ogni padre e ogni madre che vede qualcun altro scegliere per il proprio figlio sente un brivido lungo la schiena. Io amo mio figlio più di chiunque al mondo e questa è una realtà inconfutabile per ogni genitore. Ogni giorno "mettiamo sulla bilancia" ciò che riteniamo sia migliore per i nostri figli e ogni giorno facciamo una scelta. Io ho liberamente scelto, assumendomi ogni responsabilità, di vaccinare mio figlio: ho scelto pensando che il rischio che correva non poteva equipararsi al beneficio che avrebbe ricevuto; ma ho scelto io. Ministro,

Signora Presidente, signor Ministro, colleghi, il decreto su un'emergenza dovrebbe unire gli italiani e dunque anche i senatori che li rappresentano e invece è accaduto il contrario: polemiche nel Paese, clima di scontro, talora anche in quest'Aula, pareri di istituzioni scientifiche messi in dubbio e altro ancora. È una situazione senza precedenti, che giustamente si è espressa anche con migliaia di messaggi e telefonate a ciascuno di noi. Tutto questo è successo e sta ancora succedendo, perché il decreto-legge

multe fino 7.500 euro e, addirittura, il rischio di perdere la potestà genitoriale, attraverso l'intervento del tribunale per i minorenni, con un provvedimento estremo, che dovrebbe essere usato solo in casi gravissimi e non certo nei confronti di genitori, che di sicuro si occupano a fondo del benessere dei propri figli. Era, insomma, un testo punitivo, che sceglieva la via repressiva, piuttosto che quella del dialogo, della trasparenza e dell'informazione scientifica. Poi è arrivata l'ormai consueta minaccia di porre la fiducia, che avrebbe tappato la bocca a tutti - maggioranza e opposizione - e avrebbe impedito miglioramenti in Aula, anche se ampiamente condivisi.

Avemmo potuto raccontare a chi condivide le intenzioni del provvedimento di aver votato contro a causa della questione di fiducia e, a chi si oppone, di aver accolto le loro istanze, ma per gli italiani, per i genitori e per i bambini non avremmo ottenuto alcunché, nessun miglioramento delle norme e neppure l'occasione per parlarne efficacemente. Abbiamo allora scelto una via più complicata, certamente meno facile per noi, ma crediamo molto più utile per il Paese, per la salute degli italiani e di tutti i bambini. Ci siamo assunti la responsabilità di chi rappresenta il popolo e deve portare i migliori risultati possibili, prima ancora che sventolare questa o quella bandiera. Abbiamo ritenuto di dover impedire due pericoli opposti. Il primo è che fosse approvata una legge, che, per la sua impostazione errata, rischiava di produrre effetti opposti a quelli desiderati. Il secondo è che un'eventuale bocciatura di questa legge

perché pensiamo che su un provvedimento così importante non si possa decidere con un solo voto a causa della questione di fiducia, specialmente quando ci sono così tante criticità e c'è così tanta attenzione nel Paese: questo naturalmente non dovrebbe valere soltanto per i vaccini, ma, purtroppo, in altri casi non è stato così.

nostri figli; ciò è confermato dalla storia italiana e da quella europea, dove malattie che facevano un numero enorme di vittime sono pressoché scomparse e la vita media è aumentata di decenni.

Attenzione, dunque, a screditare questa pratica. Noi rispettiamo anche chi è del tutto contrario ai vaccini, ma attenzione a diffondere paure ingiustificate tra la grande maggioranza di persone che, vaccinando se stesse e i propri figli, proteggono anche coloro che non possono o non vogliono farlo. Tuttavia, così come era scritto, il provvedimento al nostro esame era ingiusto per molti aspetti e controproducente. Ci siamo confrontati allora con le associazioni dei genitori, abbiamo ascoltato le loro ragioni, abbiamo lavorato, fatto proposte, discusso a lungo e ottenuto molto, anche se non tutto quello che avremmo voluto. Abbiamo ottenuto di cambiare l'impostazione prevalentemente sanzionatoria presente in origine, per cui oggi con il testo che stiamo per approvare, prima di comminare una qualsiasi sanzione c'è l'obbligo da parte dell'ASL di convocare la famiglia, di spiegare le ragioni della vaccinazione, di fornire i dati scientifici e, solo dopo, valutare le possibili sanzioni. Tutto questo è stato fatto con un emendamento votato all'unanimità che con l'apposizione della fiducia non sarebbe stato neppure preso in considerazione.

Abbiamo fatto ricomprendere nel perimetro dell'obbligo anche i minori stranieri non accompagnati che, con un aumento degli obblighi vaccinali, era bene nominare specificamente, anche perché privi di persone per loro responsabili da assoggettare alle sanzioni.

Non è comprensibile infatti che si obblighino tutte le famiglie italiane a vaccinare i propri figli e poi non si sappia nemmeno se l'insegnante o il pediatra con cui vengono in contatto possa rappresentare un veicolo di contagio. è stato insomma profondamente modificato, dando molte risposte ai dubbi degli italiani. Rimangono però degli aspetti che ci convincono poco. Prima di tutto si sta scaricando sulle aziende sanitarie un peso enorme: centinaia di migliaia di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, da vaccinare in tempi brevissimi, senza prevedere alcun aiuto e alcun ulteriore finanziamento. Diciamo quindi subito noi abbiamo chiesto un rinvio delle scadenze, dell'entrata in vigore effettiva dell'obbligo, prevedendo per un primo periodo soltanto una forte raccomandazione e la raccolta dei dati. Avete voluto mantenere un testo dove l'obbligo è pressoché immediato. Sappiamo che già oggi le Regioni e le ASL, specialmente alcune, hanno difficoltà

evitando che l'elasticità del calendario vaccinale venisse determinata dall'incapacità e dall'impossibilità dell'ASL di mettere in atto quanto la legge prevede. Vorrei sottolineare un aspetto; la copertura vaccinale in Italia non è sufficiente e sta scendendo costantemente negli ultimi anni; lo stesso calo si verifica sia nelle vaccinazioni obbligatorie sia in quelle non obbligatorie. Non sarebbe stato meglio allora iniziare almeno tre anni fa, quando si registrava il primo calo di copertura a preoccuparsi seriamente e a controllare che la filiera della vaccinazione funzionasse, in misura maggiore sull'informazione e la conoscenza, anziché intervenire tardivamente basandosi sulle sanzioni e la repressione? Noi non escludiamo perciò e, anzi, auspichiamo ulteriori modifiche nei prossimi mesi alla luce delle difficoltà pratiche nell'attuare parti del decreto-legge. Auspichiamo che siano messi pienamente in atto aspetti che ordini del giorno ed emendamenti e hanno introdotto con riferimento alla necessità di un'adeguata raccolta delle reazioni avverse, all'attenzione dei pediatri nel valutare situazioni particolari che suggeriscono di posporre la vaccinazione (ad esempio, nel caso di bambini prematuri o, comunque, sottopeso). concludo con una considerazione di carattere generale. Il Senato, pur in una situazione di fretta eccessiva, ha dimostrato di saper fare ancora il proprio lavoro, cioè dare spazio e voce nel provvedimento alle varie opinioni e sensibilità presenti nel popolo italiano. C'è stato qualche problema, anche procedurale, forse perché si è un po' persa l'abitudine di fare il nostro lavoro e, cioè, elaborare le leggi anche attraverso momenti di scontro e di dialogo. Questa è una risposta a chi vorrebbe annichilire il Parlamento misurandone l'efficacia dalla rapidità con cui mette in atto decisioni prese altrove e che con varie campagne, che vediamo in atto da anni e anche in questi giorni, cerca di ridurne ulteriormente la portata. Con tutti i suoi limiti e difetti, il Parlamento è l'unico luogo dove le opinioni dei cittadini hanno il loro peso diretto nelle decisioni che coinvolgono tutti. Forza Italia rivendica di aver reso possibile questa discussione, di aver fortemente migliorato il provvedimento ponendo le premesse per una migliore copertura vaccinale a beneficio di tutti, anche dei non vaccinati, riducendo in modo decisivo il peso su coloro che fanno scelte diverse. Per questo Forza Italia voterà a favore di questo provvedimento.

non è la prima volta che in questa Assemblea ci troviamo ad affrontare un tema importante, il rapporto tra natura e cultura. Basti per tutti il caso Stamina, che ha visto in questa Aula momenti di grande pericolo, sventato grazie a un lavoro approfondito di conoscenza e di analisi e ad un ritorno indietro rispetto alle decisioni prese. La nascita della scienza della medicina moderna ha chiarito le strutture interpretative di questo rapporto. Non c'è natura che possa sostituirsi al progresso scientifico, a meno che a meno che non si voglia fermare la ricerca. Questo forse qualcuno lo vuole o, addirittura, si vuole vietare di mettere gli occhiali perché sono una protesi contro natura. pensiamo a cosa è successo da quando Jenner ha fatto la prima vaccinazione e a cosa succedeva prima, ci rendiamo conto che prima - lo dico a una senatrice intervenuta dicendo cose stravaganti

che ha rimesso a posto le cose e ha fatto in modo che la sicurezza dei vaccini migliorasse decisamente di giorno in giorno e di secolo in secolo. Oggi possiamo dire che le vaccinazioni sono enormemente più sicure anche solo rispetto a dieci anni fa. trovo assurda l'affermazione - sbagliata e grave - che in questo decreto-legge si faccia una sperimentazione sui bambini. È una cosa gravissima quella che è stata detta: non c'è alcuna sperimentazione. I vaccini sono sicuri e sperimentati nel mondo

un'affermazione: «L'immunità di gregge, cara signora, è smentita dalla comunità scientifica». Ma quale comunità scientifica? Quella di Wakefield? Quella che ha raccontato che i vaccini portano l'autismo? Quella è la comunità scientifica? È l'amico suo dietro casa? È qualcuno che prende soldi perché i vaccini non vadano avanti? Chiediamocelo. Avete letto tutti che oggi l'Organizzazione mondiale della sanità lancia un nuovo allarme sull'Italia, un ulteriore richiamo che fa seguito a quello dell'Unione europea

Tutti siamo stati bambini; notoriamente si cresce e se ci fossimo vaccinati prima queste cose non sarebbero successe. Passando all'obbligatorietà,

ma vorrei solo dire che dal 1999 ad oggi è cambiato il mondo e la medicina si deve adeguare ai cambiamenti del mondo. La scienza serve a questo: a parlare del mondo come è oggi, non come piacerebbe a noi o come era ieri. allora alla globalizzazione e ai contatti che si sono moltiplicati, ma non solo ai migranti perché anche i ricchi piangono e anche i ricchi portano le malattie, non so se è chiaro, lo dico a chi pensa che il problema sia solo la vaccinazione dei migranti.

tra intervento dello Stato e sfera individuale. In un mondo così deregolato i punti di riferimento sono fondamentali, perché ci orientano nelle scelte. I vaccini, allora, sono sicuri. I dati dell'Aifa sono molto chiari: nessuno dei decessi segnalati nel biennio e che si sono verificati in relazione temporale con una vaccinazione sono risultati correlati al vaccino sospettato. È chiaro? Non c'è alcuna relazione. I vaccini vanno fatti e vanno fatti nella prima fase della vita. I vaccini tutelano la salute collettiva: non basta dire «mio figlio», perché il destino è comune e la responsabilità è collettiva Quando la libertà di non vaccinarsi lede quella di chi non vuole essere contagiato, allora l'obbligatorietà è assolutamente l'unica scelta possibile. I vaccini devono tornare a essere obbligatori. Gli adulti di oggi sono stati bambini ieri e certo non possiamo aspettare i cambiamenti delle politiche industriali: dobbiamo agire ora.

Primo: diversa modulazione dell'obbligatorietà e coinvolgimento delle Regioni. A questo proposito, mi permetto di dire che il Veneto non è proprio a posto:

potenziamento della farmacosorveglianza, in modo netto e rigido. Tre: abbassamento delle sanzioni. Quattro: eliminazione del ricorso alla sottrazione della patria potestà. istituzione dell'Anagrafe vaccinale nazionale. Sei: gare anche per i monocomponenti e loro utilizzo solo nei casi certificati di immunizzazione avvenuta per le altre malattie presenti nei vaccini combinati. Sette: attenzione al diritto alla salute dei minori non accompagnati.

gli Uffici, per un lavoro difficilissimo svolto con abnegazione. Un bell'esempio di dovere civile e morale, anche per chi non era d'accordo, perché siamo andati avanti insieme e insieme abbiamo condotto in porto questo provvedimento. Coltivare il dubbio aiuta a razionalizzare le paure e a deliberare in modo informato, ma coltivare il sospetto è un'altra cosa dal coltivare il dubbio è decidere che tutto è marcio e che dietro ogni scelta c'è un interesse occulto; così viene meno il rispetto reciproco. Nella storia abbiamo perfino avuto in Italia lo spione di caseggiato, che andava, vedeva come viveva la gente e poi diceva «secondo me quello lì fa quella cosa», senza prove e senza niente. E allora, se le prove ci sono, ci sono le sedi opportune, c'è la procura della Repubblica, ci sono le sedi istituzionali e i sindacati ispettivi. Ma non si vengano però ad agitare sospetti, oltre alle nefandezze che sono state dette sui *social*. Siamo gente perbene; noi del PD siamo gente perbene!

Parliamo a tutte le famiglie, non solo a quelle famiglie le cui paure sono usate da chi è contrario alle vaccinazioni. Vogliamo

Vigileremo sull'informazione, sulla formazione, sui controlli e sull'attuazione, con le linee guida che saranno emanate dai Ministeri competenti. Se brucia la casa del mio vicino, dice un proverbio africano, la cosa mi interessa: questo è il principio della salute nel mondo globale, quello del destino comune dell'umanità.

suo decreto-legge è assolutamente incostituzionale e non sono io a dirlo, ma saranno schiere di avvocati agguerriti contro questo decreto-legge, che faranno ricorso alla Corte costituzionale e saranno appoggiati dalla NHF NHF svedese, che si occupa della difesa dei diritti dell'uomo. Ho menzionato la Svezia perché la Glaxo è stata cacciata dalla Svezia proprio per violazione dei diritti dell'uomo, perché voleva applicare esperimenti pilota sul tema vaccinale, ma è stata prontamente cacciata dal Ministro della sanità

senatore Scilipoti

Detto questo, voglio fare una riflessione e la voglio consegnare a tutti i colleghi, spiegando qual è il nostro rimprovero. Visto che noi compriamo dei prodotti e li paghiamo per averli di alta qualità e sicuri, chiedevamo che all'interno dei vaccini non ci fossero alcune sostanze additive: conservanti, particelle, nanoparticelle ed altre sostanze che potrebbero creare danni ai nostri figli. Cosa costa al Ministro che si impegnerà affinché i prodotti siano di alta qualità e che non contengano sostanze che potrebbero danneggiare la salute dei cittadini?

Signora Presidente, ribadisco che ho condiviso l'intervento del nostro capogruppo Lucio Malan nella dichiarazione di voto perché ha fatto un'analisi corretta per quanto riguarda la storia di questo decreto-legge. Viste le grandi criticità che sono già emerse nella discussione in Commissione, mi sorprende che gli stessi emendamenti presentati in Commissione da parte del Gruppo di Forza Italia siano stati respinti e che solo successivamente vi sia stata la disponibilità a considerarli. Fermo restando il fatto che noi siamo favorevoli a condividere ed a convincere le persone e non ad obbligarle, mi sorprende il fatto che il rappresentante del PD rivendichi il ruolo di questo Parlamento nella discussione; peccato che questo Governo

di tempo non potremo dire niente, ma voi avete la logica dei numeri e noi dobbiamo sottostarvi. Io consegno alla Presidenza uno studio fatto al microscopio elettronico a raggi X con relativa spettrometria, di cui ho già fatto omaggio a qualche medico che io stimo essere persona di scienza.

donna di scienza e sa bene che con la microscopia elettronica a raggi X e la spettrometria non si sbaglia. Un giorno qualcuno vi rinfaccerà che siete stati ignoranti e tracotanti al tempo stesso, perché le nanoparticelle...

Ad essi si dovrebbe fare ricorso solo in caso di stretta necessità. Qui, invece, abbiamo esagerato. In secondo luogo, non una parola e non un euro sono stati dedicati a rafforzare i servizi vaccinali: questo vuol dire non avere a cuore il funzionamento del servizio. Vorrei una sanità pubblica che fosse rispettosa del diritto dei cittadini di non essere trattati da sudditi che obbediscono in modo acritico.

ma per essere preciso. Sono venuto in Aula con tanto rispetto per ascoltare le motivazioni, perché, da genitore e da nonno, dovevo continuare a vaccinare anche i nipoti, avendo già vaccinato i figli.

Contestualmente, una parte della maggioranza ha ribadito, con argomentazioni che non mi hanno convinto, che tutti i bambini non vaccinati potenzialmente potessero causare un'epidemia...

Presidente, il mio voto sicuramente non è in totale dissenso con quanto ha detto il senatore Malan. Il mio voto è in dissenso, perché considero questo provvedimento difficilmente applicabile stante la carenza di risorse destinate alle Regioni che dovranno poi applicare le norme e soprattutto alle ASL, nonché per quel settore scolastico che sicuramente avrà difficoltà ad attuare questo decreto-legge. È troppo facile scaricare verso le Regioni, le ASL e le scuole ciò che questo decreto non contiene, ovvero le risorse sufficienti perché venga applicato. Per il resto, lo sanno tutti che sono a favore delle vaccinazioni, dunque il mio sarà un non voto.

Prima di procedere alla votazione finale, avverto che è stata presentata ed è in distribuzione una proposta di coordinamento presentata dalla relatrice, che si intende illustrata. *(Commenti del senatore

possano realmente capire cosa state votando e lo chiedo anche per i colleghi del PD.

«All'articolo 1: a) al comma 4: 1) al primo periodo, introdotto dall'emendamento 1.110 (testo3), sostituire le parole: «gli affidatari» con le seguenti: «i soggetti affidatari»; 2) al secondo periodo, come modificato dagli emendamenti 1.110 (testo 3), 1.116 e 1.112 (testo 3), sopprimere le parole: «e alla persona cui il minore sia stato affidato» e sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-*bis*»; 3) al terzo periodo, sostituire le parole: «di cui al primo periodo» con le seguenti: «di cui al secondo periodo»; b) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Disposizioni in materia di vaccini». *All'articolo 5, alla rubrica, aggiungere infine le parole:* «e finali»

deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione,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 Nel corso della seduta di ieri la 1a Commissione permanente ha espresso parere favorevole sulla sussistenza dei predetti presupposti e requisiti. Successivamente, da parte del prescritto numero di senatori, è stato richiesto su tale parere il voto dell'Assemblea. Domando all'estensore del parere, senatore Maran, se intende intervenire.

Ci troviamo di fronte a un decreto-legge che viola almeno una trentina di norme della Costituzione, tra cui norme di diritto tributario, civile e fallimentare, nonché le direttive europee in tema di concorrenza. arriviamo a vedere la consegna di fatto del monopolio del credito di un'intera Regione strategica per l'economia nazionale, quale il Veneto. Andiamo a consegnare di fatto il credito a un'unica banca, ottenendo in regalo quasi nuovi 900 sportelli e un insieme di strutture dell'istituto di credito, nonché un patrimonio di tipo anche edilizio.

all'inizio quella norma, assolutamente irresponsabile, che ha imposto l'obbligo della quotazione in borsa per le banche popolari, tra cui Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, ha provocato il primo tracollo di un patrimonio tracollo di un patrimonio per una Regione dove le imprese investivano e c'era la possibilità di avere finanziamenti. Stiamo parlando di un mondo di risparmiatori e azionisti che hanno purtroppo investito in azioni, trovandosi oggi perfettamente truffati. Ci troviamo di fronte a persone che hanno creduto a dirigenti e funzionari

separati in base al diverso titolo di credito che vantano nei confronti della banca. Non solo: c'è una disparità di trattamento anche rispetto a coloro che sono stati

sembrava che le banche popolari venete fossero al riparo da tutti i rischi. Quella che di queste banche veniva data era un'immagine avvalorata da mezzi di comunicazione, certificata da organi di controllo interni ed esterni e avvalorata persino dalle procure,

con la responsabilità di Banca d'Italia, Consob e di tutti coloro che dovevano intervenire e controllare. Ma quello che qui è venuto a mancare è proprio il principio di giustizia, perché il Governo in questi anni non ha fatto il minimo sforzo, non ha intrapreso alcuna azione per ristabilire quel senso di giustizia che viene chiesto dai risparmiatori e dagli azionisti, non essendo stati né individuati né puniti i responsabili. E la giustizia è stata negata ai risparmiatori soci, i quali si sono visti vittime sacrificali di operazioni elaborate sopra la loro testa. Hanno perso i risparmi di una vita. Hanno perso anche la possibilità di avere un sostegno per la vecchiaia e la malattia e ora, con la privazione dei diritti, hanno perso anche la dignità. Noi ci siamo attivati per sostenere che questo provvedimento non si deve fare e che, comunque, è illegittimo sotto il profilo costituzionale. Noi continueremo a insistere - abbiamo proposto le nostre iniziative, che saranno contenute anche in quella mozione di cui chiederemo la discussione - affinché siano inasprite le pene per chi commette dei reati a livello dirigenziale all'interno delle banche: per la truffa, l'aggiotaggio, le false comunicazioni, l'ostacolo all'esercizio delle funzioni e della vigilanza. Negli Stati Uniti, il signor Zonin sarebbe già andato in galera. Noi qui abbiamo delle fattispecie di reato irrisorie. Vogliamo che all'azione di responsabilità debba conseguire anche l'interdizione perpetua dell'esercizio delle professioni e soprattutto degli uffici direttivi, in particolare di impresa e istituti bancari. Vogliamo che sia prevista l'ipotesi di bancarotta fraudolenta anche per questi soggetti, che ne diverranno quindi imputabili. Vogliamo che sia aumentata la platea dei risparmiatori ammessi alle procedure di ristoro.

è come vedere attualizzati ad oggi i valori dei danni che subimmo durante la guerra. Abbiamo gli stessi identici valori. È stata messa in ginocchio una popolazione che ha grande dignità e che continuerà a lavorare.

questo Paese non uscirà dall'emergenza finché la classe politica, eletta in Parlamento con leggi elettorali a suo uso e consumo, vive, prospera e lucra sulle emergenze. Nelle emergenze riesce a imporre ogni sua bassezza, ogni grottesca decisione al popolo. Le emergenze sono il cavallo di Troia per qualsiasi furberia, come - ad esempio - regalare due banche al prezzo di un euro al primo gruppo bancario italiano e garantirgli che in questa operazione sia lo Stato, cioè i cittadini, a coprire costi e rischi. Ma quale affare? Risarcire i risparmiatori: questa era una misura urgente. Miliardi, invece, si sono volatilizzati e vengono sottratti all'economia del Veneto e del Nord-Est. Avete lasciato morire i consumatori, i risparmiatori e adesso scaricate i costi di un salvataggio tardivo sui contribuenti. Ve lo dico in Veneto: *vergogneve*! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Nessuno vuole lasciare i lavoratori in mezzo a una strada, ma questo vale anche per tante altre realtà produttive ignorate invece dal Governo. Nessuno vuole che, dopo migliaia di risparmiatori, anche i correntisti siano travolti, ma la soluzione era un'altra: nazionalizzare. Se deve essere lo Stato a mettere le risorse per risanarle, poteva e doveva essere lo Stato a ricavarne i frutti. Due banche pubbliche in Veneto, con una *governance* ripulita, avrebbero svolto la funzione di far ripartire il credito alle famiglie, stimolando i consumi, e verso le imprese sane, strozzate dal *credit crunch*: questa era una misura urgente. Quello che emerge dalle inchieste è che lorsignori prestavano soldi facili a politici, come i 7,5 milioni dati a Verdini per pagare le sanzioni per le irregolarità del Credito cooperativo che non erano - per così dire - solvibili, dalla vecchia Alitalia all'Acqua Marcia di Francesco Bellavista Caltagirone, e siamo ancora in attesa di avere la lista completa di tutti i soggetti. Sarebbe davvero illuminante. A volte questo avveniva contro il parere stesso dei tecnici della banca. Intanto, i clienti senza santi in paradiso, per avere credito, erano indotti ad acquistare azioni di una banca che stava diventando un colabrodo. Inchiodare le responsabilità: questa era una misura urgente. Invece siete riusciti a bocciare la calendarizzazione urgente della nostra mozione in merito. E grosse responsabilità hanno anche i colleghi veneti del PD: mi riferisco ai senatori Santini, Filippin, Dalla Zuanna e Puppato. I cittadini devono sapere che, con questo decreto, implicitamente si aiutano i responsabili a farla franca, perché, se a fronte di un fallimento che è già nei fatti, i responsabili fossero verosimilmente perseguiti per bancarotta fraudolenta, i limiti di prescrizione si innalzerebbero, e forse avremo la speranza di vedere conclusi i processi. Così invece è gravemente probabile la prescrizione. Quella contro la prescrizione è la madre di tutte le battaglie. Il Movimento 5 Stelle esige che, dopo una condanna in primo grado, i cittadini abbiano garanzia che giustizia sia fatta. Voi scommettete sull'intasamento della giustizia per garantire l'impunità. dal Gruppo M5S)*. Voi dovete sapere che niente come l'impunità stimola nuovo malaffare e nuova corruzione. Le procure sono allo stremo: Treviso è terzultima nel rapporto giudici-cittadini. Mancano quattro giudici e due sostituti. Il ministro Orlando dice che non ci sono carenze. Ma anche la Lega ha le sue responsabilità. Cosa ha fatto? Governava Treviso, la Regione e aveva il ministro della giustizia Castelli. I responsabili della devastazione economica del Nord-Est resteranno impuniti se non verranno date risorse aggiuntive. Serve un *pool* straordinario: questa è una misura urgente. Abbiamo a che fare non con un terremoto improvviso, ma con un'agonia che dura da quasi dieci anni. La crisi bancaria mondiale è nota dal 2008. Altri Governi, di economie ben più solide, sono intervenuti massicciamente: 400 miliardi di dollari di interventi diretti e indiretti ai crediti considerati a rischio del sistema bancario furono disposti immediatamente da George W. Bush. Nel Regno Unito furono stanziati 50 miliardi di sterline di investimento di Stato e 41 miliardi chiese la Spagna al Fondo salva-Stati, finanziato anche da noi italiani, peraltro a debito. La Germania è intervenuta con la bellezza di 197 miliardi tra aumenti di capitale e titoli tossici rilevati dallo Stato federale e dai *Länder*: una cifra - sono dati della Commissione europea - che vale il 7 per cento del PIL tedesco. Mentre il disastro era sotto gli occhi di tutti e tutti gli Stati riconoscevano il pericolo, in Italia si parlava come segue. Il 10 ottobre 2008, Berlusconi diceva: «l'Italia ha il sistema bancario più solido di Europa». Pochi giorni dopo, Bersani spiegava Bersani spiegava che l'Italia aveva il sistema bancario più solido, perché c'era stata una buona vigilanza da parte della Banca d'Italia e aggiungeva anche che, per quanto potesse risultare amaro, ciò era merito pure di Fazio, così come adesso è merito di Draghi. 7 ottobre 2011, Fabrizio Saccomanni, direttore generale di Banca d'Italia, dichiarava: «Gli istituti di credito hanno un grado di solidità e di capitalizzazione assolutamente adeguato in relazione agli *standard* europei». Nel gennaio 2012, Mario Monti, Presidente del Consiglio, diceva: «Il sistema bancario italiano è tra quelli più stabili sulla comparazione internazionale». 5 agosto 2013 Enrico letta, Presidente del Consiglio, affermava: «La ripresa è vicina e il sistema bancario italiano è solido». Nell'aprile 2014, Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, davanti all'assemblea dei soci di Veneto Banca, interveniva sui controlli già scarsi e tardivi di Bankitalia: «Quello della Banca d'Italia a Veneto Banca è stato un attacco senza precedenti alla nostra identità e alla nostra autonomia che fa parte di un disegno contro tutte le banche territoriali, popolari e Bcc che siano. Da oggi la battaglia si fa sempre più dura ed è un bene che Consoli sia rimasto». Il 29 dicembre 2015 non poteva mancare "il bomba", Matteo Renzi, il quale ha dichiarato che «il sistema bancario italiano è solido» e «non lo cambierei con quello tedesco». Tutto l'arco parlamentare, ma potrei dire del partito unico, che possiamo riconoscere nelle sciagurate parole di Piero Fassino - «Abbiamo una banca» - ha tenuto il prosciutto sugli occhi e levato il pane di bocca ai veneti. Intervenire solamente qualche anno fa avrebbe consentito di limitare i danni. Mentre la politica ballava sul Titanic, le banche hanno visto invece la fuga dei correntisti, peggiorando le condizioni. E il tessuto economico veneto ha subìto conseguenze drammatiche che, a livello macro, richiederanno sacrifici enormi, mentre a livello dei singoli, delle singole aziende e delle famiglie, sono saltati progetti di vita e la vita stessa è finita per sempre. Appare dunque evidente che i requisiti di necessità e urgenza, anche ove sussistenti, sono conseguenza di inerzia, omertà e incompetenza, se non di cinico calcolo, giacché oggi assistiamo a un'accelerazione improvvisa che consente un patto patto diretto con un soggetto privato, senza le dovute garanzie di trasparenza, e uno spreco di risorse pubbliche. Si tratta di un decreto-legge che regala a Banca Intesa oltre 5 miliardi di euro per tenere invariati i propri livelli di patrimonio e altri 12 miliardi di euro di

non può essere meramente enunciata in modo apodittico, ma deve ravvisarsi nel contenuto del provvedimento. si può considerare doveroso intervenire, dall'altro dobbiamo denunciare che questa situazione si è venuta a creare non già per un terremoto, ma per colpa del Governo e degli organi di controllo, che la soluzione proposta lascia totalmente scoperte le principali priorità, i diritti dei risparmiatori - ciò a beffa dell'articolo 47 della Costituzione - e i diritti dei cittadini di avere giustizia di avere giustizia e di vedere ben utilizzate le risorse pubbliche. Il decreto-legge arriva blindato e verrà posta la fiducia su un testo inaccettabile e offensivo. Non abbiamo alcuna possibilità che le necessità e le urgenze vere del Paese siano alla fine rispettate. Il Movimento 5 Stelle, dunque, ritiene non sussistano i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione. Signor Presidente, come Sinistra italiana ieri in Commissione abbiamo votato contro i presupposti di necessità e urgenza del

alla concorrenza Margrethe Vestager, a margine di un vertice con il Governo italiano, svelò alcuni retroscena molto sorprendenti

un eventuale salvataggio delle due banche da parte del Governo avrebbe costituito una zavorra sul consenso.

un bel regalo, senza mai porsi il problema dell'istituzione di una vera banca pubblica a sostegno di una politica creditizia a favore degli investimenti, in particolare delle piccole e medie imprese.

tramite un comunicato ufficiale, che l'operazione non avesse alcun impatto sul proprio patrimonio e sulla sua politica di distribuzione dei dividendi e che, comunque, l'esito

nel senso che, se vi azzardate a fare alcune modifiche che a noi non sono gradite, il contratto viene dichiarato nullo. Credo che nella storia della Repubblica non si sia mai verificata una cosa simile. Non parliamo poi - sempre dal punto di vista della

Signor Presidente, giunge nell'Aula del Senato un decreto-legge che mostra una fotografia impietosa di quanto accaduto negli ultimi anni al sistema bancario italiano all'economia italiana e, in particolare, a quelle banche che, essendo più vicine all'economia reale italiana che sta sui territori, che compone il nostro modello di industrializzazione, e cioè la piccola e media impresa, hanno sofferto di più

quando guardiamo alle valutazioni dell'Europa, dobbiamo sempre ricordarci che quell'Europa ha stabilito di rispondere alla crisi finanziaria in atto nel pianeta nel modo forse peggiore e, cioè, nascondendo la capacità di quelle banche della cooperazione

il combinato disposto della crisi e delle valutazioni dell'Unione europea, la quale, per annullare il rischio, impone criteri di patrimonializzazione così alti da mettere in difficoltà il nostro sistema bancario, che è fatto di banche grandi, medie e piccole, cioè di una differenza e di una concorrenza che hanno sempre garantito al nostro Paese il migliore utilizzo della leva finanziaria nello sviluppo e nel sostegno delle imprese. Questo è il contesto nel quale dobbiamo calare la nostra valutazione

stato urgente, come avete detto tutti (e lo si poteva collocare, pur nell'ambito di quelle regole europee che puntavano a cancellare le peculiarità italiane, a metterle in difficoltà,

una percentuale davvero minima nel sistema bancario italiano) e di Monte dei Paschi di Siena, che invece costituiva una forza rilevante nei numeri del sistema bancario italiano,

Tutti e tre questi grandi casi sono stati affrontati in modo completamente diverso: qualche volta d'accordo con l'Unione europea in cambio di qualcos'altro, altre volte invece subendo, come nel caso di Banca Etruria, il peggiore dei trattamenti.

una peculiarità alla quale ancora non avevamo mai assistito. Noi potevamo nazionalizzare quelle banche, e non solo quelle venete; potevamo partecipare a quelle banche, come ha fatto per esempio il Governo tedesco con le sue; potevamo garantire la concorrenza del mercato, e cioè la libera concorrenza tra i privati. i privati. Nel caso delle banche venete al danno si aggiunge la beffa, perché qualche altro investitore istituzionale privato, oggetto peraltro della recente riforma delle banche di credito cooperativo, aveva sì avanzato una proposta per risolvere la questione, mantenendo così quella caratteristica peculiare di vicinanza al territorio e al sistema delle piccole e medie imprese che a tutti noi sta a cuore. Tuttavia, ciò è stato impedito

socializza tutte le perdite e garantisce la privatizzazione di quegli utili che ci saranno - e Dio sa quanti ce ne saranno una sola banca, in omaggio a quella visione europea che noi contrastiamo, per cui il sistema bancario deve essere fatto da due o tre grandi banche, mentre invece va cancellata ogni traccia di polverizzazione sul territorio, che considero un elemento che favorisce la concorrenza e ha aiutato il sistema delle imprese a sopravvivere anche negli anni più duri della crisi. Del resto, se non ci fossero state quelle banche, non credo sarebbe esistito il modello Nord-Est; se non ci fossero state quelle banche nelle Marche, l'impresa e l'economia di quella Regione sarebbero state quelle che sono diventate? No, niente affatto. allora io vorrei domandare al Governo se non si rende conto, sottosegretario Baretta, che per la prima volta introduciamo un'innovazione legislativa: una fiducia obbligatoria che, invece di votarla al Governo nel rispetto delle regole democratiche di questo Paese, votiamo a una banca. Perché quella banca si è permessa di scrivere - e voi avete accettato questa condizione - che nessuna modifica di quel testo avrebbe potuto essere accettata da Banca Intesa. E allora la prossima volta le leggi fatevele fare da Banca Intesa!

è un totale oltraggio agli articoli 1 e 47 della Costituzione. In base a tale provvedimento, dovrebbero essere i risparmiatori e i lavoratori a pagare per una dirigenza scellerata, per enormi prestiti concessi senza alcuna garanzia. condanna migliaia di piccoli e medi risparmiatori, infatti, a vedersi togliere ogni possibile speranza di far valere le loro ragioni, a fronte di documentate e criminali azioni volte ad ingannarli. Questa storia non riguarda investitori professionisti o speculatori, ma persone semplici e risparmi di famiglia. Riguarda i lavoratori e i piccoli e medi imprenditori, che sono sempre stati il cuore pulsante della Regione Veneto, che si sono suicidati o che hanno tentato di farlo; riguarda tutti coloro che avevano fatto affidamento su quei risparmi per assicurare una vita dignitosa ai propri figli, dopo anni di duro lavoro; riguarda tutte le imprese fallite e tutti coloro che avevano un posto garantito grazie a quelle stesse imprese. E, infine, riguarda tutti coloro che rischiano di perdere la propria casa. Qualche giorno fa l'Ecofin, il Consiglio europeo dell'economia e delle finanze, ha deciso che ogni singolo Stato dovrà istituire una *bad bank*, dentro la quale dovranno confluire tutti i crediti inesigibili delle banche, i famosi NPL, così come accadrà anche per le due banche venete. Confedercontribuenti Veneto, però, ha già analizzato oltre 4.000 che più di 3.000 di questi sono contestabili per diversi illeciti e vizi contrattuali e contabili. Questo è l'ennesimo schizofrenico provvedimento che ci sta imponendo l'Europa, con la piena e incondizionata collaborazione del nostro Governo, che regala decine di miliardi alle banche, lasciando nella disperazione migliaia di famiglie e aziende.

e più di 800.000 occupati, per la maggior parte in aziende di piccole dimensioni. Il settore è in crisi perché i prezzi dei prodotti agricoli (frutta e verdura) sono in calo da anni,

deduco che i due Gruppi parlamentari non abbiano ancora designato i senatori che dovrebbero far parte di tale Commissione e con la loro condotta continuano, fino a questo momento, ad impedire che la Commissione sia già operativa. Mi rivolgo, anche in questo caso, direttamente alla Presidenza: sarebbe importante sapere quali sono i due Gruppi che non vogliono che si faccia chiarezza, attraverso una Commissione d'inchiesta, sulle vicende relative alla ricostruzione dell'Aquila. Alcune fonti di stampa nazionali e locali, proprio ieri, hanno annunciato 10 nuovi arresti e 35 nuovi indagati per gli appalti postsisma. Tra questi, funzionari pubblici, professionisti, imprenditori ed alcuni rappresentanti del Segretariato regionale del Ministero dei beni culturali e della Soprintendenza

partire. Ricordo ancora una volta alla Presidenza che la Commissione d'inchiesta è stata deliberata da questa Assemblea il 10 novembre scorso, con l'approvazione del relativo documento a mia prima firma. Da allora, è trascorso un lasso di tempo molto ampio che avrebbe permesso di svolgere un lavoro

faccia presto il suo dovere, nominando la Commissione d'inchiesta sull'Aquila. Per quello che riguarda l'atto vandalico, se ne stanno già occupando il comandante provinciale e i Carabinieri dell'Aquila.